L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi martedì scorso, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea. Nella giornata odierna sarà esaminato il decreto-legge in materia di stabilizzazione finanziaria. La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 19 luglio, l'Assemblea esaminerà i disegni di legge recanti l'istituzione della Commissione diritti umani, la nuova disciplina

Oggi è possibile dire ragionevolmente che l'Italia, nonostante lo scenario dell'ultima settimana (il riferimento è alle Borse), è uscita dalla crisi in condizioni comparativamente migliori, non si è fatto ricorso, come si chiedeva da più parti, a manovre di stimolo fiscale, che avrebbero aggravato i problemi, in quanto, com'è noto ai più, non si sarebbe potuta contrastare la recessione globale con un'azione anticiclica nazionale. Il deciso rifinanziamento degli stabilizzatori automatici, segnatamente degli ammortizzatori sociali, ha consentito comunque di fornire un sostegno a coloro che sono stati investiti dalla crisi in prima persona. Nel frattempo, la crisi greca e quella di altri Paesi europei in difficoltà di finanziamento dei loro debiti sovrani hanno reso ancora più instabili i mercati finanziari, e ciò si riflette sulle remunerazioni richieste per il finanziamento di tutti i debiti stessi. Gli attacchi speculativi, che non si manifestavano prima della crisi globale, oggi sono molto più difficili da controllare, e ne abbiamo avuto una prova evidentissima nei giorni scorsi. I mercati finanziari valutano più che in passato i debiti nazionali in base alla crescita economica che ne garantisce la sostenibilità a lungo termine. Nel 2010 siamo usciti della recessione sempre con un basso tasso di crescita, ma più vicini a quello medio europeo, se si fa l'eccezione della Germania. La nostra casa non brucia, ma la guardia deve essere tenuta molto alta. Ciò significa che in termini dinamici la sostenibilità della nostra finanza pubblica è oggi più elevata di quella della gran parte dei Paesi europei. L'impegno dell'Italia è quello di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014. Proprio in sede europea, il piano italiano è stato valutato e apprezzato. Per gli anni 2011 e 2012 gli obiettivi posti sono garantiti sostanzialmente dai provvedimenti già adottati. La combinazione della manovra al nostro esame, così come rafforzata dal pacchetto di emendamenti che ho inteso proporre durante l'esame in Commissione, che si è concluso nelle prime ore di questa giornata (alle 3,30 di questa mattina), punta a garantire il piano di azzeramento del deficit nel corso del biennio successivo. In questo contesto, la riforma della *governance* in ambito di Unione europea, approvata di recente, ha prodotto un importante rafforzamento delle regole a presidio della sana gestione delle finanze pubbliche dei Paesi che ne fanno parte, formulando un innovativo *iter* procedurale che realizza un legame tra riforme da attuarsi, nel senso di un rafforzamento delle economie e dell'innalzamento del livello di competitività, e la disciplina e il controllo delle finanze pubbliche. Quanto alla manovra, con riferimento agli 2011 e 2012, le variazioni di spesa e di gettito tendono a compensarsi e ad avere un impatto trascurabile sui saldi tendenziali. I maggiori effetti di contenimento si concentrano negli anni 2013 e 2014, riflettendo le indicazioni programmatiche previste dal Documento di economia e finanza approvato in quest'Aula ad inizio aprile. Sulla base delle stime, che sono riepilogate nel provvedimento, la manovra netta in termini di indebitamento prima delle modifiche in Commissione aveva un effetto di 17 miliardi sul 2013 e 25 miliardi sul 2014. La composizione della manovra per il 2011 anche se di impatto trascurabile sui saldi, è caratterizzata da un aumento netto delle spese e delle entrate. In particolare, in termini di indebitamento, nel primo esercizio nel primo esercizio le spese e le entrate aumentano di circa 1,8 miliardi rispettivamente, mentre nel 2012 la variazione è pari a oltre 4 miliardi. La composizione della manovra per gli anni 2013 e 2014 evidenzia sia un aumento netto del gettito fiscale, rispettivamente di 7 e 6,6 miliardi, sia una riduzione netta delle spese per circa 11 e 19 miliardi. Per effetto degli emendamenti approvati in Commissione, i saldi migliorano ulteriormente di oltre 2 miliardi nell'anno corrente, circa 5 nel 2012, 6 nel 2013 e 22 nel 2014. Appare pertanto non pienamente condivisibile la presunta intenzione di rinviare il risanamento, in quanto sull'anno in corso e quello a venire agiscono già, come è ovvio, i dispositivi contenuti nei provvedimenti pluriennali approvati in precedenza: i decreti-legge n. 112 del 2008, n. 78 del 2009 Nei primi tre anni di Governo sono stati infatti operate consistenti correzioni in una fase congiunturale nettamente peggiore di quella che stiamo vivendo. Il punto dolente, semmai (e lo dico come parlamentare e non come relatore), è indagare i motivi della loro non compiuta realizzazione, per i motivi più diversi, tutti meritevoli di approfondimento tecnico

Ma il pareggio di bilancio non costituisce l'unico obiettivo da assicurare per evitare rischi di instabilità, non essendo in secondo piano anche l'obiettivo di innalzare il tasso di crescita dell'economia del Paese, che al momento si profila per i prossimi anni assai limitato. Si rende dunque necessario, nel delineare un percorso di correzione strutturale della finanza pubblica, nel senso del perseguimento di un permanente riequilibrio tra la dinamica della spesa e quella delle entrate, l'intervento di azioni correttive incisive sui macroaggregati della spesa, non disgiunte da misure che tendano a migliorare l'andamento del denominatore, ossia elevino il tasso di crescita Il risultato di contenimento della spesa già conseguito nel 2010 è stato sicuramente positivo, perché, per la prima volta dopo decenni, la spesa primaria è scesa in valore assoluto, segnando una flessione di 14 miliardi rispetto a quanto previsto dal Governo. In tal senso, appare oggi indispensabile l'attivazione di tagli di spesa «selettivi», come suggerito dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, a partire dalla spesa delle amministrazioni pubbliche per i consumi intermedi, che è stata pari nello scorso esercizio a 136,1 miliardi, anche se in leggera flessione rispetto al 2009. Nel complesso, è chiaro che, al fine di pervenire alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa, occorre partire da una lotta senza agli sprechi, su cui potrà senz'altro avere un ruolo di peso il metodo sistematico della *spending review*, anzitutto per le amministrazioni centrali, i Ministeri, così come delineato nello schema di decreto attuativo della legge di contabilità. In questo quadro, la manovra di aggiustamento del bilancio pubblico e il disegno di legge di delega della riforma fiscale rappresentano, presi congiuntamente, un passaggio cruciale, non solo per l'azione di governo, ma per il futuro del nostro Paese, per il futuro dell'Italia.

Il capitolo sui costi degli apparati politici apporta un correzione in gran parte prudenzialmente non cifrata ma di sicura rilevanza. Il capitolo della razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche comprende una decisa riduzione delle spese dei Ministeri. In tema di acquisti di acquisti di beni e servizi, si adottano interventi per la razionalizzazione dei relativi processi di approvvigionamento individuando misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti tramite la CONSIP. In tema di operazioni di acquisto e vendita di immobili, segnalo la previsione di procedure di verifica preventiva del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia. grazie a tutti vigili sulle Casse di previdenza privatizzate attribuendole il controllo sugli investimenti delle relative risorse finanziarie. In tema di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, sono previste l'estensione al 2014 del blocco degli stipendi pubblici già prevista dall'ultima manovra triennale e la proroga delle disposizioni limitative delle assunzioni. In tema di spesa sanitaria, è contemplato un intervento in materia di beni e servizi: l'Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento al fine di mettere a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio

In materia previdenziale, è prevista la progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quelli delle lavoratrici del settore pubblico, anche se con tempi molto graduali. altresì una misura finalizzata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pensionistica del biennio 2012-2013, sopprimendo l'indicizzazione delle fasce alte di importo, superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, poi, con azioni emendative, anche con un contributo di solidarietà per importi di pensione per importi di pensione superiori ai 90.000 e ai 150.000 euro. In tema di Patto di stabilità interno, si dispone il concorso alla manovra delle Regioni a statuto speciale, delle Regioni a statuto ordinario, Tali interventi sono assistiti da previsioni di nullità dei contratti di servizio in contrasto ovvero elusivi delle regole del Patto di stabilità interno e da sanzioni nel caso di violazione del medesimo. In materia di entrate, sono previste, tra l'altro, la tassazione separata sull'attività di *trading*, ovvero sulle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria, l'aumento dell'imposta di bollo sui depositi titoli, così come l'applicazione dell'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie. Si introduce, a partire dal 2011, una addizionale annuale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 kilowatt. capitolo in tema di riorganizzazione del processo civile, con una serie di interventi che portano a una semplificazione, a uno snellimento e a una velocizzazione delle procedure. Lo sviluppo non è assente dal provvedimento. Il titolo secondo è interamente dedicato al tema, con misure di agevolazione della contrattazione aziendale, un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e in mobilità, la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e la liberalizzazione del collocamento, con la completa attuazione della legge n. 30 del 2003 (legge Biagi).

Presidente, colleghi, il provvedimento esce notevolmente rafforzato dall'esame della Commissione. Si è inteso altresì rispondere con una celere approvazione ai segnali che il mercato ha manifestato nei giorni scorsi. In merito a ciò, c'è una grande prova di responsabilità e dignità - non so se spetti al relatore questa considerazione - del Parlamento italiano, al di là delle diverse opinioni anche sulle misure di intervento. La risposta

ascoltato durante le audizioni. È stata una prova di grande democrazia. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i colleghi

Gentile, Giorgetti e Casero, e naturalmente il presidente Azzollini che fino a poche ore ha governato e portato a conclusione l*'iter* del provvedimento, con una serie di azioni di cambiamento. Sono stati pochi ma qualificatissimi gli emendamenti per qualità e quantità materiale, finanziaria, non numerica. Un primo emendamento è diretto ad anticipare la ripresa di efficacia delle norme in materia di quote di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (*ticket*). Una seconda modifica interviene sulle misure in materia previdenziale, in particolare - ed è quella cui accennavo prima - rivedendo in senso migliorativo il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni di importo inferiore a cinque volte il minimo (nel senso che inizialmente il provvedimento era peggiorativo, rispetto alla condizione attuale, per le pensioni di più basso importo)

la tempistica per l'esercizio associato di funzioni da parte di enti locali e vengono meno le riduzioni di risorse a favore degli enti locali. Infatti, è stata ricostituita una parte del fondo del fondo di perequazione. È stata poi rivista la disciplina dell'imposta di bollo sui *dossier* titoli rimodulando gli importi dell'imposta in considerazione dell'ammontare del deposito titoli.

L'emendamento di maggiore portata finanziaria comporta una riduzione dell'accantonamento destinato al fondo per gli interventi strutturali di politica economica e rende definitivi gli accantonamenti già disposti già disposti dalla legge finanziaria per il corrente anno in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle aste per le frequenze. Si dispone infine che i regimi di esclusione ed esenzione fiscale, di cui all'allegato

Si tratta di una misura di evidente e rilevantissima portata, finalizzata a ricondurre entro i limiti del pareggio di bilancio nel 2014 i conti pubblici, anticipando in sostanza uno dei principali contenuti della delega fiscale già approvata dal Consiglio dei ministri. Mi sia consentito di concludere queste note sottolineando come l'adozione di una articolata gamma di interventi che vada nel senso di una riduzione della spesa, senza intaccare i livelli di servizio della pubblica amministrazione, presuppone, prima di ogni altra cosa, che si abbia chiara l'urgenza del momento e l'indifferibilità delle misure di risanamento. È un'azione che può salvare il patrimonio degli italiani che lo hanno, ma garantire anche lo Stato sociale, tanto necessario a coloro che il patrimonio non ce l'hanno. Nei giorni scorsi abbiamo toccato con mano gli effetti dei segnali che un rafforzamento della manovra e una accelerazione del suo *iter* può avere sulla fiducia dei mercati. Ciò impone una visione politica che guardi lontano, oltre gli interessi immediati e particolari delle singole componenti sociali e comunità locali, che sia ispirata dalla capacità di scegliere e guidare per rendere possibile ciò che è giusto, ciò che è doveroso, ciò che è necessario alla qualità della vita umana. Taluni hanno detto, non senza ragione, che la recessione è stata paradossalmente una benedizione per l'Italia, perché, causando un brusco arretramento assoluto, ne ha acuito il bisogno di cambiamento e l'ha reso non più procrastinabile. La riduzione della pressione fiscale deve essere accompagnata e preceduta dalla riduzione della pressione regolamentare, per liberare l'innovazione, nel settore privato come nel settore pubblico. La riforma fiscale è strategica, in questa prospettiva, non perché essa possa comportare nell'immediato una riduzione complessiva della pressione fiscale, ma perché determini una profonda modifica strutturale del prelievo che rifletta la rottura degli interessi corporativi. Questo stesso spirito deve guidare la riduzione della spesa pubblica, necessaria a ottenere il pareggio di bilancio senza aumento delle tasse. Una riduzione della spesa che deve avere origine dall'aumento che deve avere origine dall'aumento dell'efficienza e da una analisi attenta delle priorità. Il problema della bassa crescita italiana, è ormai chiaro a tutti, così come il malessere della società, sta, prima di ogni altra cosa, essenzialmente in un mancato raccordo tra la domanda di beni e servizi,

La lenta crescita, la lunga perdita di competitività, le buste paga ferme e i profitti bassi di oggi sono tutti indicatori che parlano chiaro alla politica: le non scelte o le riforme solo parziali hanno sinora avuto l'unico esito di bloccare l'economia e la società, con un danno reale per tutto il Paese nel suo insieme. Perché l'Italia torni a crescere è dunque indispensabile superare definitivamente una fase di assuefazione alle condizioni di lenta crescita registrata negli ultimi anni, dal momento che non ci si accorge che stando fermi, in realtà, si arretra rispetto alle altre economie e al reddito che si sarebbe potuto generare, mancando in tal modo una preziosa opportunità per noi e per le generazioni future. *(Applausi

2814** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci eravamo illusi che l'atto di grande responsabilità delle opposizioni, in un momento così drammatico per il nostro Paese, potesse mutare gli orientamenti del Governo sulla politica economica e di bilancio. Pensavamo, questo sì, che potesse svilupparsi un confronto su aspetti limitati del provvedimento, quelli che avevamo sottoposto al Ministro dell'economia nella giornata di martedì, incontrando la sua attenzione e disponibilità. Così non è stato. Alle tre di questa notte abbiamo concluso i lavori in Commissione con risultati molto deludenti. Può tale chiusura al confronto, di cui parlerò più diffusamente in prosieguo, rimettere in discussione la nostra importante decisione politica di consentire un esame velocissimo di questo provvedimento? No, non è avvenuto in Commissione e non avverrà in Aula, perché la ragione del nostro atteggiamento non risiedeva dentro lo spazio di una trattativa, che non c'è mai stata, ma era ancorata all'appello del Capo dello Stato e all'estrema gravità della situazione che si era determinata e che voglio qui brevemente ripercorrere. Il giorno della presentazione della manovra correttiva al Senato è il 6 luglio; la Borsa di Milano ha chiuso in forte calo, a meno 2,44 per cento, dopo una seduta segnata da difficoltà in tutta Europa. Il giorno dopo, giovedì 7 luglio,

evidentemente anche la notizia che la manovra presentata dal Parlamento ha una dimensione macroeconomica effettiva inferiore per almeno 15 miliardi rispetto a quella annunciata

tra i titoli italiani e tedeschi raggiunge il record storico di 305 punti e Piazza affari sprofonda del 3,96 per cento, con una perdita di capitalizzazione di altri 16 miliardi. È quella la giornata dell'appello del Capo dello Stato alla coesione nazionale, subito responsabilmente accolto dalle opposizioni, secondo

per affrontare e superare le difficili prove che già sono all'ordine del giorno». La giornata di martedì, infatti, in seguito alle decisioni politiche cui mi sono riferito, dopo dopo un primissimo segnale di panico nella prima mattinata, riporta la calma nei mercati e le contrattazioni in equilibrio. La sintetica cronaca degli eventi accaduti nei mercati finanziari spiega più di ogni altra considerazione tattica e politicistica la posizione assunta dalle opposizioni in Italia: consentire di approvare la manovra più pesante della storia repubblicana, dopo quella del Governo Amato del 1992, in tempi rapidissimi, come mai prima si era verificato, in modo da porre un argine al baratro che si era aperto. D'altronde, nelle giornate di lunedì e martedì gli appelli, le sollecitazioni e le prese di posizione erano stati univoci: «Fate in fretta, mettete in sicurezza il Paese»; lo avevano detto il Presidente della Repubblica, l'Eurogruppo e le parti sociali tutte. Le opposizioni, nella persone dei presidenti dei Gruppi Finocchiaro, Belisario e D'Alia, nella giornata di lunedì hanno anticipato il Governo, chiedendo formalmente al Presidente del Senato di anticipare i lavori d'Aula per consentire di concluderli oggi, e lo stesso sforzo hanno fatto i Gruppi e la Presidenza della Camera; solo dopo è pervenuta una nota scritta del Presidente del Consiglio, il grande assente di questa cruciale fase storica, preso com'è dai suoi problemi e dalla sua irrimediabile debolezza politica. L'altro ieri il Ministro dell'economia ha ringraziato le opposizioni, con un gesto sincero che abbiamo apprezzato (anche perché insolito, come ha dichiarato la nostra presidente espressivo della gravità di questo passaggio della storia del nostro Paese. Voglio sottolineare questo passaggio. Le opposizioni, anche un solo Gruppo, anche pochi senatori, avrebbero avuto tutti gli strumenti regolamentari, e non mi riferisco neanche a quelli ostruzionistici, per chiedere un normale andamento, differendo i lavori di fatto di una o due settimane. Così non è stato, la politica questa volta ha fatto la sua parte, almeno per quel che riguarda il tema della tempestività della decisione pubblica che si imponeva. L'opposizione, e il nostro Gruppo in particolare, non è stata presente soltanto nei momenti drammatici che ho ricordato. Siamo stati presenti e vigili in tutti questi tre anni, denunciando l'inadeguatezza della vostra politica economica e finanziaria, aggravamento dei fondamenti della nostra economia e della finanza pubblica, mentre il *mantra* era che l'Italia aveva reagito meglio degli altri, che la finanza pubblica era stata risanata, che i conti erano sotto controllo e così via. È fin troppo facile constatare che così non era e non è. era e non è. Ma il nostro Gruppo nei mesi scorsi, in parallelo all'*iter* di approvazione progressiva della riforma della *governance* economica europea, ha più volte richiamato l'attenzione del Senato italiano a discutere approfonditamente e per tempo il Piano nazionale delle riforme, non solo perché l'Europa ce lo imponeva, ma soprattutto per la necessità di avviare le riforme strutturali invocate da circa 15 anni e mai realizzate. E c'eravamo quando abbiamo discusso il DEF ad aprile.

2011 di fronte ad un Governo tentennante che stentava a dichiarare ciò che era evidente, ovvero la necessità di agire subito e per tempo. Questo ed altro proponevamo agli inizi di maggio. La Commissione europea, lo scorso mese di giugno, ha formulato la sua raccomandazione e ha detto all'Italia esattamente ciò che era già stato detto dal nostro Gruppo

e forse - nessuno di noi può affermarlo con certezza, ma certo il dato cronologico fa sorgere fondati dubbi sul punto - vi è una relazione tra l'incompletezza e l'incertezza del contenuto della manovra e ciò che è accaduto nei mercati in questi giorni. Dunque, nel Parlamento italiano non c'è una maggioranza che vuole il risanamento e un'opposizione che non la vuole, semmai è vero il contrario per tutto ciò che ho appena detto. Il nostro giudizio di inadeguatezza e scarsa credibilità dell'intervento correttivo proposto si basa soprattutto, lo abbiamo detto dall'inizio, sulla totale assenza di adeguate e convincenti misure per sostenere la crescita della nostra economia. Non c'è alcun dubbio che la manovra determinerà effetti negativi sulla crescita dell'economia. Come ha detto il Governatore della Banca d'Italia il 31 maggio scorso nelle sue considerazioni finali, e ha ribadito ieri, in Commissione bilancio, vice direttore della Banca d'Italia, ci sarà un effetto depressivo sul PIL di due punti percentuali. La crescita doveva essere sostenuta dal Piano nazionale delle riforme e dal decreto sviluppo, ma è a tutti evidente che ciò non si verificherà. Dunque, la grande assente della politica economica dell'Italia è una seria strategia per la crescita e la credibilità della manovra di bilancio è gravemente minata da tale debolezza. Lo dicono tutti: le organizzazioni le organizzazioni sociali, datoriali, sindacali, i commentatori di ogni orientamento politico; ce lo ha ricordato il professor Mario Monti in un articolo del 3 luglio scorso e nuovamente questa mattina sul "Corriere della Sera". Il 3 luglio il professor Monti sottolineava che poco o niente viene fatto per immettere più concorrenza nel settore dei servizi, nelle industrie a rete, nelle professioni. C'eravamo illusi, nella giornata dell'altro ieri, quando il ministro Tremonti aveva annunciato un'incisiva misura di liberalizzazione e privatizzazione. Invece, all'esito, supponiamo, dello sbarramento di componenti importanti della maggioranza, la norma che solo ieri è stata depositata costituisce un virtuosismo normativo e politico che dimostra in modo inequivocabile che il freno a mano continua ad essere tirato da braccia molto forti. Il Governo, secondo la norma che avete approvato, decide di proporre

Noi abbiamo presentato un pacchetto serio, credibile e immediatamente efficace di liberalizzazione, naturalmente respinto, come avete fatto numerose volte in questi tre anni. Signora Presidente, abbiamo preso atto positivamente che il Governo si è fatto carico di integrare la manovra fino all'importo concordato in sede europea. Lo avevamo chiesto per le ragioni cui ho accennato all'inizio Ci era sembrato che allo sforzo di concentrazione temporale e contenutistico che avevamo promosso e che abbiamo puntualmente operato, seguisse una naturale apertura al confronto corso del rapidissimo esame del provvedimento in Commissione. Invece non è andata così. Avete blindato, anche in questo circostanza, un testo che aveva amplissimi margini di modifiche e miglioramenti, a saldi invariati. Dunque, il nostro giudizio negativo non muta, anzi per taluni aspetti si aggrava, perché era a portata di mano la possibilità di fare di più e meglio.

a tentare di superare le sue divisioni e contraddizioni e il Governo ingessato e incapace di interloquire. Nessuna parola è stata spesa né dal Governo, né dalla maggioranza, per mezzo del suo relatore, sulle serie e credibili proposte emendative delle opposizioni.

un pacchetto serio, e non una presa in giro, sui costi della politica con l'anticipo al 2012 dell'equiparazione del trattamento economico dei parlamentari a quello dei Paesi di testa dell'area euro; dei parlamentari per superare l'insostenibile sistema attuale sostituendolo con quello contributivo. Sì, lo abbiamo scritto, proposto

l'inclusione dei *referendum* nell'*election day;* la proposta di una sola società pubblica per ciascun Comune; l'introduzione di un tetto ragionevole alle retribuzioni dei dirigenti pubblici e l'accorpamento delle Province. Anche al riguardo l'opposizione,

Voto contrario della maggioranza (PdL e Lega) su tutto. Nessuno di questi argomenti è stato preso in considerazione. Avevamo chiesto di ripristinare trasparenza e concorrenza Avevamo chiesto di ripristinare trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici eliminando la norma estensiva (e scandalosa) della trattativa privata per lavori fino a 1 milione di euro (il 96 per cento degli appalti), le norme note sui grandi eventi (quelli della «cricca»), la segretazione degli appalti SOGEI, di cui si discute in questi giorni. Nonostante l'assenso di massima del Ministro su tali argomenti, non vi è stata neanche una parvenza di interlocuzione. Avevamo chiesto di rivedere la norma sui *ticket* introducendo, quanto meno, robuste soglie di esenzione basate sull'ISEE, e invece le avete anticipate. Da domani i poveracci, i deboli, le famiglie, i pensionati, i lavoratori saranno costretti, per vostra scelta, a pagare *ticket* PD*). Avevamo chiesto di rivedere la riduzione del fondo sanitario nazionale e del patto di stabilità interno e invece avete prodotto un ulteriore ed incomprensibile pasticcio targato Lega (la norma sul patto di stabilità è incomprensibile ed inattuabile sotto il segno della virtuosità). Avevamo chiesto di eliminare alcune marchette, come si dice in gergo parlamentare,

i medici e gli infermieri. Vi avevamo chiesto di rivedere i pasticciati interventi sull'ICE, che rischia di paralizzare qualunque sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e sull'ANAS. tolte alcune limitate modifiche alla riforma del processo del lavoro e agli interventi iniqui su pensioni, patrimoniale sui titoli e ammortamenti (peraltro, con soluzioni pasticciate con aumenti dell'IRAP e così via),

La credibilità della manovra è ciò che più ci preoccupa e che rischia di riattivare la speculazione - speriamo di no - vanificando i sacrifici che state chiedendo al Paese. Si può, signori del Governo e della maggioranza, pensare seriamente di ottenere un contributo al risanamento nella misura enorme di 20 miliardi di euro da un disegno di legge delega sulla riforma fiscale e sull'assistenza, il cui contenuto è richiamato nel decreto ed è tuttora ignoto al Parlamento e al Paese? No, non è serio pensarlo. Delle due l'una: la riforma fiscale non sarà fatta, nel qual caso - lo prevede la norma - a pagare saranno soltanto, ancora una volta, i ceti più deboli, cioè beneficiari delle prestazioni sociali, delle detrazioni e delle deduzioni fiscali che si vogliono tagliare del 15 per cento (notoriamente i redditi alti non usufruiscono in modo significativo di deduzioni e detrazioni), oppure la riforma si farà; poiché non è pensabile di ricavare dal capitolo assistenza (pensioni sociali, indennità di accompagnamento e poco altro) una cifra al 10 per cento dei 20 miliardi previsti nella manovra, si determinerà un drastico aumento della pressione fiscale. Dunque, state nuovamente elevando in misura consistente la pressione fiscale. Il

di quasi due punti percentuali: altro che la favola della riduzione delle tasse che state raccontando al Paese da anni, su cui vi siete accapigliati, avete litigato in questi giorni all'interno del Governo e della maggioranza! Con questo decreto state decidendo di aumentare le tasse di

Il ministro Padoa-Schioppa nel 2007 disegnò il percorso della *spending review*, introducendolo nel nostro sistema contabilistico pubblico. contabilistico pubblico. Voi lo avete dolosamente abbandonato in questi 3 anni, reintroducendolo in modo blando in questa manovra. Vi abbiamo chiesto di accrescere il peso della riduzione degli sprechi e dei costi dell'apparato pubblico - e non il peso delle entrate fiscali - fissando le regole fissando le regole della revisione della spesa, alla quale non avete mai creduto e mostrate di non credere. Se anche nel passato, nel primo anno di avvio, esse non davano ancora - per ovvi motivi - risultati questo non significa negare che quella è la vera via per mettere mano ad una seria, costante, stabile riduzione «La qualità di un'idea si rivela dalla sua capacità di rinascere dai propri insuccessi», disse il compianto ministro Padoa-Schioppa, citando Altiero Spinelli, nel giugno del 2007. Noi vi abbiamo fornito i testi (lo ha fatto in modo efficace e testardo il collega Morando) di una nuova *spending review*, dell'introduzione della regola del pareggio del bilancio e dei modi per conseguirlo nella legge di contabilità. Anche queste proposte sono state respinte, senza spendere una parola e senza alcuna interlocuzione. Pensavamo, signora Presidente, che la paura, purtroppo purtroppo fondata, e la lezione di questi giorni potessero rideterminare un clima di unità del Paese assimilabile a quello vissuto, pur in un contesto molto diverso, con il Governo

temiamo, sperando di sbagliarci, che non sarà Sufficiente, e che il cammino da qui al 2014 sia ancora lungo e fangoso. Ci siamo battuti per migliorarla e continueremo a farlo, ma ce lo avete impedito. Il clima di responsabilità e fiducia che abbiamo contribuito a determinare è stato decisivo per i mercati e per l'Europa. C'è un altro messaggio che urge: quello di porre fine a questa vostra esperienza di Governo e di dare al nostro Paese un nuovo Governo all'altezza della terribile sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni. anni. Questo sarà l'argomento all'ordine del giorno a partire da dopodomani.

di almeno mezz'ora, per definire alcuni adempimenti che sono legati alla manovra, anche perché ritengo che possano essere presenti persone importanti e responsabili del Paese che potrebbero dare delle risposte più dettagliate rispetto alle questioni che abbiamo sollevato in questi giorni.

la Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Pertanto, conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

la 5a Commissione si è riunita e prima di tutto ha dovuto prendere atto che, innovando seppur di poco una prassi che si va consolidando nel Senato, il testo della Commissione ha subito delle variazioni: una in diminuzione e due in aumento.

proprio con questa Presidenza si era introdotta una modifica in positivo, e ciò mi pare da rimarcare; e speriamo che continui. l'impianto complessivo della manovra è quello uscito dalla Commissione bilancio; in particolare, tutti gli emendamenti di rilievo approvati sono regolarmente e identicamente contenuti nel testo sul quale il Governo ha chiesto la fiducia.

alla sua unanimità e il Governo l'hanno ritenuta coperta regolarmente, qualche perplessità è stata manifestata da parte dei colleghi dell'opposizione sull'innovazione di cui all'articolo 27. I colleghi dell'opposizione hanno ritenuto di rinvenire nella suddetta norma dei profili di scopertura, in particolare con riguardo al suo estendersi

la norma manca di copertura, e dunque andrebbe espunta. Il Governo ha risposto con due puntuali argomentazioni. Per quel che riguarda

del periodo di vigore dell'agevolazione. Su tutto il resto, la Commissione ha convenuto. Presidente, sono un po' perplesso dall'*incipit* dell'intervento del presidente Azzollini, il quale ha dichiarato

due soltanto. Rispetto al passato, quando abbiamo assistito a ben altra percentuale di innovazioni - che non mi permetto di ricordare a tutti voi perché avete vissuto con me la storia di questo Parlamento - credo si possa registrare con positività da parte di questa Presidenza aver innovato e aver voluto fortemente, così come continuerà a volere fortemente, che qualora una Commissione esiti un testo per l'Aula ed il Governo decida di porre la fiducia, la fiducia venga posta sul testo della Commissione. Abbiamo fatto passi in avanti grazie a tutti noi, e io continuo a essere vigile.

noi siamo arrivati numerosissime volte ad espungere dal testo su cui era stata apposta la questione di fiducia importanti parti del testo scelto dal Governo, perché il tema non era stato affrontato e non era stato discusso e votato dalla Commissione. quindi vero che stiamo applicando adesso questo principio sulla base di un maggiore rigore di quanto non sia accaduto in passato. Stiamo applicando lo stesso rigore e, dato il clima politico che si era e si è determinato, di collaborazione sul punto che riguarda la rapidità con cui affrontare il passaggio del Senato su questa manovra, mi auguravo che in questo caso il Governo rispettasse al 100 per cento l'impegno che si era preso a non modificare il testo uscito dalla Commissione. Credo che il Governo avrebbe fatto meglio a comportarsi così, così, anche in omaggio alla collaborazione che gli è venuta dall'opposizione. Detto questo, però, la seconda modificazione di cui stiamo parlando, signor Presidente, non è affatto marginale, e riguarda un aspetto molto rilevante, su cui attiro l'attenzione del Ministro dell'economia in particolare. Noi abbiamo, signor Presidente, all'articolo 27, una norma che, sostituendo ciò ciò che nel gergo veniva chiamato forfettone per aziende marginali - che sono 600.000 in Italia - afferma un regime speciale di tipo fiscale con aliquota al 5 per cento per nuove imprese. Non si discute qui ovviamente il merito della scelta, ma la norma originaria, non modificata in Commissione, prevede che questo regime speciale al 5 per cento - quindi un'agevolazione fortissima si applichi per l'anno d'imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi. L'emendamento,

grazie alla limitazione a quattro esercizi successivi a quello in cui avviene l'inizio dell'attività di impresa, è del tutto evidente che, se prevedo che si applichi un'aliquota al 5 per cento per gli anni successivi al quarto, si determina un problema di scopertura finanziaria.

Ora, lasciamo perdere il merito, ma dove sta scritto che questa limitazione a 35 anni è in grado di compensare la possibilità di andare oltre i quattro anni di cui parlava il decreto originario? Assolutamente da nessuna parte. Il Governo non ha presentato corretta relazione tecnica,

Signor Presidente, signori senatori, il decreto oggi in votazione ha data 6 luglio. La crisi finanziaria, iniziata nel mondo cinque anni fa, si è radicalizzata in Europa a partire dall'autunno del 2009, traendo origine dalla Grecia, ed è esplosa pochi giorni fa. L'economia greca è pari a solo circa il 3 per cento dell'economia europea, ma ha un rilievo sintomatico e sistemico che la trascende. Siamo dentro un paradosso: l'area dell'euro è oggettivamente l'area più ricca e meno indebitata del mondo e, tuttavia, la percezione che oggi ne hanno i mercati finanziari non riflette questa forza. Anzi, a giudicare dal valore dei CDS, dentro la classifica dei Paesi valutati come i più rischiosi al mondo, ai primi tre posti ci sono tre Paesi dell'area dell'euro. Ovviamente, ciascuno di questi Paesi (Grecia, Irlanda e Portogallo) ha importanti problemi da risolvere, ma la scala relativa è assolutamente fuori da ogni logica. A giudicare dagli *spread* dei titoli sovrani sui titoli tedeschi, oggi i mercati finanziari ritengono ad alto rischio investimenti in un'area pari al 40 per cento del PIL dell'Unione monetaria. Nessuno ci può credere, ma è proprio questo il problema. Più che di speculazione finanziaria, è un problema di credibilità e di fiducia politica: perché credere in una moneta fatta da 17 diversi Stati-Nazione, governata da 17 diversi Governi controllati da 17 diversi Parlamenti? Nella storia, prima viene lo Stato e poi viene la moneta. Con l'euro si è invertito l'ordine: prima la moneta e poi, solo in prospettiva, l'Europa federale. I trattati internazionali sono costruiti come i matrimoni: di norma sono contratti nella buona e nella cattiva sorte. Non così i trattati di unione: qui il bene è la regola, il male solo l'eccezione. La crisi finanziaria si aggira per il mondo come un mutante, che oggi appunto prende la forma della Grecia. Diceva Churchill: «I Balcani e la Grecia producono più storia di quella che consumano e per questo la esportano». È così che oggi abbiamo in Europa un appuntamento con il nostro destino. La salvezza non ci viene dalla finanza, può venire solo dalla politica; ma la politica non deve più fare errori. Non possiamo dire prima, a Bruxelles in primavera, che in Europa tutto, tutti i titoli recanti le nostre firme sovrane, sono garantiti, e poi dopo, a Deauville in autunno, dire che tutto può invece essere perso. È così che ora siamo arrivati insieme al dilemma e al dramma dell'euro e dell'Europa: o si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è; o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic, non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Non è solo una questione specifica di singoli Stati: è una questione comune che riguarda la credibilità politica dell'euro e dell'Europa. Serve una visione alta sul nostro futuro, serve la costruzione di una *governance,* capace di guidare unitariamente ed autorevolmente i 17 Paesi membri verso un destino comune. La logica politica che da sempre è parte della costruzione europea, la logica di risolvere i problemi interni dei Paesi membri per facilitare il processo di unione, si è come ribaltata. In alcuni Paesi sembra che si antepongano i problemi interni alla costruzione comune. L'estrema destra della destra sta dando in molti Parlamenti un contributo negativo in questo senso. Nel 2003 ho riproposto l'idea degli eurobond. Ne ho poi scritto con il Primo ministro del Lussemburgo, Presidente dell'Eurogruppo. Credo, con molti altri, che questa idea - finora non abbastanza sostenuta - sia comunque l'idea giusta. Italia: non ci può essere una politica italiana diversa da quella europea, e viceversa. L'impegno per il pareggio di bilancio è stato preso in Europa, e in Europa è stato preso dall'Italia il 27 marzo scorso. È così che siamo arrivati a questo decreto, rafforzato in questi giorni. Dalla Commissione europea, dall'OCSE, dalla Germania sono venute valutazioni positive sulla nostra manovra: valutazioni positive che sono in parte sfuggite in Italia. L'aggravarsi della crisi ha reso, se non era sufficiente, ancora più evidente la ragione politica di questo decreto: un decreto che non è solo di finanza pubblica. Questo decreto, sommato al decreto sviluppo appena convertito, oltre alle azioni già fatte negli anni passati, contiene 16 nuove azioni per la crescita: azioni che vanno dal credito d'imposta per la ricerca alla detassazione dei nuovi contratti di produttività, dalle imprese dei giovani al credito d'imposta per il Sud, dal processo civile al turismo, dalle zone a burocrazia zero alle reti di impresa e ai fondi d'impresa, dalle opere pubbliche alle ristrutturazioni private in casa propria, dalle privatizzazioni alle liberalizzazioni. Vedete, il bilancio pubblico lo si fa tutto per legge. Il PIL non si fa solo per legge. Servono, certo, decreti come questi, e come altri. E si può fare di più. Sentiremo tutti su tutto, ma non si può dire che dal lato dello sviluppo non è stato fatto niente finora. Davvero non è corretto. E in ogni caso, senza la tenuta del bilancio pubblico, con i suoi effetti sociali ed economici, non ci sarebbe neppure stato il PIL che c'è stato finora. Ciò che serve ora è un duro, responsabile lavoro comune, nel Paese, per il Paese. Ma torniamo al bilancio pubblico. La manovra di finanza pubblica è esatta e corretta ed allineata sull'asse del tempo, esattamente come concordato in Europa. Nessuno ci chiede di fare il pareggio di bilancio nel 2011. Ma tutto impone di definire già dal 2011 l'intero percorso per arrivare al pareggio di bilancio nel 2014, così costituendo da subito un vincolo assoluto al pareggio: un vincolo insieme giuridico e politico. Il nostro lavoro non termina oggi. Dovremo insieme - insieme maggioranza e opposizione - introdurre nella nostra Costituzione la regola d'oro del pareggio di bilancio. Concludo. In aggiunta a quelle molto forti fatte finora, nessuno fa una manovra come questa, peraltro, se non perché vuole il bene comune. Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e dei nostri figli. Il Paese ci guarda: guarda il Governo, guarda la maggioranza e guarda l'opposizione, certamente diversi, ma oggi qui non troppo divisi. Per questo sono orgoglioso di essere qui oggi con tutti voi.

di apprezzamento per il lavoro svolto in questi giorni in tempi immediati per dare una risposta ad una speculazione finanziaria che ha toccato gli interessi economici del nostro Paese. Non posso sottrarmi da un ringraziamento specifico al senso di responsabilità del Governo, che è stato tempestivo nel formulare proposte innovative,

Questa è una risposta forte, ispirata al principio della solidarietà istituzionale e della coesione nazionale cui ci richiama sempre, quasi quotidianamente, il nostro Presidente della Repubblica. Sarei felice se momenti come questi, non dietro la spinta di un'emergenza ma dietro la quotidianità della politica, si potessero ripetere, in una logica di confronto e di rispetto reciproco, in maniera tale che la politica dell'ascolto, cui mi richiamo sempre, possa trovare piena attuazione, nelle Commissioni e in Assemblea. Credo che faremmo un servizio al Paese e daremmo un senso di sicurezza delle nostre istituzioni ai cittadini, che ce lo chiedono quotidianamente.

signori del Governo, colleghi, credo di dovere un ringraziamento al Ministro per l'approccio che ha avuto rispetto al dibattito, al confronto e per l'impostazione della sua relazione. Il ringraziamento è anche una valutazione positiva rispetto a quanto emerso durante il dibattito che ha preceduto questo incontro, questa riunione, questa occasione e questa circostanza di oggi. oggi. In realtà, quello che è emerso, prima ancora del merito del confronto e del dibattito, è una risposta di carattere politico: maggioranza e opposizione hanno recuperato, in un sussulto di comune responsabilità, una capacità di dialogo e confronto, che significa la risposta della politica ad un'esigenza politica e ad una questione politica. Ringrazio il Ministro, perché l'approccio che volevo dare all'intervento a nome del Gruppo che, tra l'altro, si chiana e si definisce di Coesione Nazionale non a caso, non era di tipo

il modo migliore per fronteggiarlo era recuperare il listino dei valori: sono emersi in questo dibattito parole, definizioni, immagini, suggestioni che richiamano alla fiducia, alla stabilità, alla coesione, all'interesse nazionale, al bene comune, cioè alla politica, alla capacità della politica d'interpretare, di rappresentare e di comunicare il servizio alla comunità nazionale dentro il grande scenario della crisi che stiamo fronteggiando. Bisogna riconoscere che il migliore interprete di questo stato d'animo, di questo sentimento e insieme di questa esigenza è stato chi rappresenta per definizione, per ruolo, per funzione e per Costituzione l'unità nazionale. cioè riconoscere che il Presidente della Repubblica ha svolto una funzione alta, nel senso più alto del valore della politica, quando ha dettato l'agenda ed i tempi ed ha

nel corso degli anni, il che consente un intervento più morbido nel 2011-2012 e più fortemente concentrato, come l'Europa richiede, nel 2013-2014. È stato il Presidente della Repubblica a interrompere questo circuito della contrapposizione schematica e di mero schieramento, strumentale rispetto agli interessi in gioco, richiamando tutti alla coesione nazionale. Quest'ultima è poi l'essenza della contrapposizione bipolare matura e della democrazia dell'alternanza come competizione tra proposte di governo e funzione governante, per chi è alla maggioranza e per chi, dall'opposizione, tende a diventare maggioranza, interpretando meglio di chi governa l'interesse nazionale, e non di parte. Abbiamo recuperato questa dimensione che dovrebbe appartenere alla normalità della politica,

grazie a tutti entro la fine di quest'anno, di impegnare 6,7 miliardi di euro e di certificare spese per 8,8 miliardi di euro, di cui 7 miliardi di euro nel Mezzogiorno, e abbiamo il dovere nazionale di individuare le scelte che consentano a questa massa enorme di risorse di diventare un investimento per la crescita. In tal senso, il nostro contributo è stato volto a far inserire nella manovra un riferimento che individua un luogo di coesione istituzionale e sociale all'interno della Conferenza Stato-Regioni, apre alle parti sociali, articolo 32, commi da 13 a 15 della manovra, al fine di individuare in essa le scelte di collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli e della funzione del sistema, per fare concentrazione delle risorse, individuazione delle opere

Anche così, nella pratica e nella capacità di governo, si danno risposte politiche all'interno della crisi. L'obiettivo che allora tutti dobbiamo auspicare, la direzione di marcia che tutti dobbiamo perseguire è quella di costruire, a partire da domani, la capacità di maggioranza e di opposizione

della modernizzazione istituzionale e della crescita economico-sociale del nostro Paese. Anche in questo caso, vorrei fare un riferimento, e poi concludo, al signor Presidente della Repubblica. Nel 2006, in occasione della Fiera del Levante, in un luogo simbolo del Mezzogiorno, il Presidente della Repubblica parlò dell'esigenza di intervenire in via sistemica rispetto agli sprechi dell'intermediazione politica, e a quella che egli definì la congestione istituzionale, come elemento fondamentale di modernizzazione e di moralizzazione del sistema. Abbiamo di fronte la grande prateria del cambiamento e del rinnovamento di questo Paese, che non appartiene al Governo Berlusconi ma all'Italia, al suo futuro, alla sua prospettiva e capacità di essere protagonista nel grande scenario globale, recuperando il dibattito

realtà, nella modernizzazione italiana, abbiamo bisogno di riflettere sulla nuova statualità. Una nuova statualità e una nuova socialità rappresentano il grande impegno che le forze politiche hanno di fronte per manifestare, al di là del ruolo e della funzione temporanea, capacità e cultura di governo. Con questo spirito e per questo obiettivo, pur nella consapevolezza che si può fare di più e meglio, riteniamo che oggi sia un dovere civico e politico sostenere il Governo e la manovra che siamo chiamati ad approvare.

né per la congiura sistemica degli gnomi della finanza, che aggrediscono in modo protervo un Paese piuttosto che un altro. Certo, è vero - come lei ci ha ricordato - che c'è un attacco all'euro e alla sua credibilità per le debolezze strutturali e le contraddizioni profonde che riguardano la moneta unica, ma se la nostra economia è stata sottoposta ad una condizione di così grave difficoltà, dietro questa azione c'è un Esecutivo che ha perso grande credibilità, che ha dimostrato, dopo tre anni, una serie di debolezze sempre più strutturali, che ha contrasti evidenti al suo interno in cui c'è lo stridore profondo di conflitti, anche personali, di grande spessore. il conflitto tra gli esiti di questa politica economica e gli annunci ottimistici, banalizzanti, che hanno caratterizzato la comunicazione politica del Governo, e in modo particolare, del Presidente del Consiglio, tutta tesa a negare la profondità della crisi, le difficoltà della nostra economia per questa idea tanto televisiva e tanto da *spot* di un Paese sereno e felice che invece si avviava verso il baratro. c'è anche il limite della sua politica economica, che non ha avuto la capacità di stimolare la crescita e che si è caratterizzata per una scelta asfittica di tagli lineari, senza una vera aggressione alle sacche di inefficienza e che, anche dal punto di vista sociale, è stata iniqua.

Senza alcun cedimento vi è stato il taglio lineare al Mezzogiorno, nel senso letterale: avete tirato una riga sotto il Garigliano e separato il destino del Paese. Non c'è mai stato in tanti anni un tale trasferimento di risorse pubbliche destinato alle politiche di coesione a favore delle aree più forti del Paese. avvenuto certamente per la cultura e l'ispirazione profonda di questo Governo che ha nel Nord il suo *core business* e nella forza di soggetti politici come la Lega, vero azionista di riferimento del Governo, ma è anche il frutto di quell'impasto strano di iniquità sociale derivante dalla vostra cultura politica, che ritiene debba prevalere sempre la legge del più forte, in una sorta di malintesa interpretazione della dottrina liberale secondo cui la competizione è selvaggia. Mentre la dottrina liberale pretende l'eguaglianza dei punti di partenza, voi la interpretate in un modo distorto e brutale in cui prevale la legge del più forte

come regola generale e astratta che garantisce i consociati. E ciò, non solo, signor Ministro, nel tanto noto caso della norma "salva-Fininvest", ma anche in casi minori e meno noti, ma non per questo meno gravi, come quello che riguarda una ferrovia locale che è stata commissariata con un provvedimento del Governo che interferisce con un procedimento giurisdizionale giurisdizionale in cui è fissata l'udienza violando in modo preciso le regole dello Stato di diritto. Non perdo certo l'occasione odierna per ricordarle questo, come ho già fatto personalmente dandole un appunto; lei mi ha ascoltato ma, come al solito, non ha fatto nulla. Questa è l'ennesima occasione perduta nel rapporto politico che c'è stato tra il nostro movimento con l'attuale coalizione e con questo Governo. A causa di tale meccanismo, in cui mancate di equità e di solidarietà, state perdendo il senso di un destino comune di questo Paese; state determinando la rottura dell'unità nazionale. In questo contesto e di fronte alla disponibilità delle opposizioni, nata per l'invito autorevolissimo del Capo dello Stato, a cui anche noi abbiamo risposto dando il nostro contribuito affinché i tempi per l'approvazione della manovra fossero brevissimi, pensavo che in seno all'esame di un provvedimento così importante vi fosse lo spazio per avviare una interlocuzione serena anche su queste vicende; che vi fosse lo spazio per dare qualche segnale di sviluppo all'economia meridionale, come elemento di stimolo e non di assistenza, come sollecitazione per far ripartire il Paese

Oggi nel Paese c'è una crisi grave, come c'è nella vostra maggioranza: il vostro disimpegno verso il Mezzogiorno, la disattenzione che mostrate in merito alle responsabilità che avete assunto nei confronti di quell'area del Paese

raccolto nelle aree meridionali, a cui anche noi abbiamo dato il nostro contributo, che si fondava su un grande piano di crescita e di sviluppo di cui il Sud stesso era parte. Ebbene, tale piano è stato tante volte annunciato, ma il processo di intervento strutturale, sistemico di sviluppo non è stato mai

Per quanto un Parlamento sia costruito intorno ad una legge elettorale che non legittima gli eletti, il successo del leadertrascina la coalizione garantendo i successi personali. tale carisma viene meno, quando la crisi avanza, anche il vostro ceto politico, quello insediato nelle Regioni meridionali, entra in gravissime difficoltà. I segni della crisi sono molto evidenti, e lei, signor Ministro, dovrà farsene carico

quindi, signor Ministro, che l'attuale maggioranza sia giunta al capolinea: è in piena contraddizione, ha fallito il suo rapporto con il Paese, ci ha dato una manovra iniqua, una risposta inaccettabile, non è stata corretta nella gestione dei rapporti tra maggioranza ed opposizione in una fase tanto delicata.

per le dichiarazioni che ha reso questa mattina in Aula, che sono sostanzialmente identiche a quelle che lui ha avuto la cortesia di rendere ieri ad una riunione privata, seppure di un'autorevolissima associazione come l'Associazione bancaria italiana; non ha avuto altrettanta cortesia a venire ieri, in tutta la giornata o questa notte, in Parlamento per spiegare il rafforzamento della manovra, cioè il motivo dell'ulteriore aggiunta di 20 miliardi di tasse. Comunque, prendo atto del fatto che questa mattina la parte sulla crisi, che abbiamo ascoltato ieri in diretta televisiva SKY, è stata ripetuta a favore della diretta televisiva RAI (probabilmente per la *par condicio*).

maggioranza ed opposizione, di voler rispettare gli impegni europei e l'azzeramento del deficit pubblico al 2014. Abbiamo promosso un ordine del giorno, insieme alle altre forze dell'opposizione, che impegna il Governo e tutte le forze politiche rappresentate nell'Aula del Senato per questa legislatura e per la prossima. Il secondo pilastro è il codice genetico progettuale e programmatico del nuovo Gruppo, l'identità politica, che poggia su un tridente: rigore finanziario, crescita economica ed equità sociale.

la nostra proposta di manovra, che non è poggiata sulla mistificazione dei tagli sugli anni futuri tendenziali, che determinano aumenti di spesa pubblica, né sull'ingiustizia dell'oppressione fiscale e dell'aumento delle entrate, ma sui tagli veri, verticali e non orizzontali, che contengono i veri costi della politica. Questo è il nostro codice genetico. A ciò si affianca la proposta di politiche per la crescita che hanno effetti di medio-lungo termine, ma che sono urgentissime. Mi riferisco alle liberalizzazioni alle privatizzazioni, a partire dalle cosiddette ex municipalizzate fino agli ordini professionali.

così come è stata presentata al Senato aveva tre difetti. Innanzi tutto, non azzerava il deficit pubblico e non rispettava gli impegni europei; luogo, l'aggiustamento era spostato quasi totalmente al 2013-2014; infine, nella sua composizione frenava l'economia e la crescita e quindi, attraverso il freno sulla crescita,

e questo, sommandosi ai 25 miliardi della manovra arrivata in Senato, adesso, aritmeticamente, *ex ante*, consente di far vedere che nel 2014 l'Italia farà deficit zero. Vengo agli altri due difetti, signor Presidente. Che cos'è questa manovra, alla luce dell'emendamento di ieri sera e anche dei piccoli aggiustamenti di questa mattina? Prendo la tabella del Ministero dell'economia e delle finanze dell'ultimo Documento di economia e finanza, sovrappongo la tabella che misura gli effetti della manovra della Ragioneria generale dello Stato ottengo i seguenti risultati. Dopo questa manovra, auspicando che venga approvata al più presto possibile - ma dobbiamo avere la consapevolezza di quel che stiamo decidendo - le entrate pubbliche passeranno dai 722 miliardi dell'anno scorso a 842 miliardi nel 2014, a dimostrazione che i tagli sui valori futuri tendenziali nascondono aumenti di spesa pubblica. La spesa complessiva passerà dai 793 miliardi del 2010 agli 842 miliardi del 2014. Ecco allora che nel 2014 avremo 842 miliardi di spesa, pari a 842 miliardi di entrate, e deficit zero. Ma cosa stiamo decidendo? Di aumentare le entrate di 120 miliardi; di usare 120 miliardi per tagliare 70 miliardi di deficit; di usare 50 miliardi di maggiori entrate e di maggiori tasse per finanziare 58 miliardi di aumenti di spesa corrente e 8 miliardi in meno di investimenti. Allora, è evidente che si produrrà un effetto di freno sulla crescita che, da questo punto di vista, può mettere in dubbio anche l'obiettivo del deficit zero. Ultimo punto, signor Presidente. Si è detto da parte del Governo che il biennio 2011-2012 è comunque tenuto sotto controllo dalla manovra precedente. È vero. Ma se l'aggiustamento è sul 2013-2014, vuol dire avere la consapevolezza che da qui al 2014 avremo, dopo la manovra, circa 140 miliardi di debito pubblico in più, che sono la somma dei 61 miliardi del 2011, dei 40 miliardi del 2012 e dei 40 miliardi del 2013. Quindi faremo deficit zero, con qualche dubbio, nel 2014, ma nel frattempo avremo accumulato 140 miliardi in più di debito pubblico che,

miliardi di interessi in più. Ecco allora che il freno sulla crescita ed il maggiore debito rischiano di mettere in dubbio lo stesso obiettivo di deficit pubblico.

Presidente, Ministro dell'economia, colleghi, dopo annunci, tensioni e scontri nella maggioranza bufera sui mercati, approda in Aula una brutta, bruttissima manovra. Si tratta di una manovra distante anni luce dall'impostazione sociale ed economica dell'Italia dei Valori, una manovra che però ci dicono potrebbe salvare il nostro Paese dal rischio *default*, vera e propria bancarotta per l'Italia. Per queste ragioni, abbiamo evitato di porre in essere manovre ostruzionistiche, che sarebbero state peraltro vanificate dal quarantaseiesimo voto di fiducia. E proprio la posizione di particolare,

credibilità che solo la fermezza e la guida autorevole del Capo dello Stato hanno evitato che venisse fatta a brandelli. È una manovra che ha impiegato più tempo per arrivare da Palazzo Chigi al Quirinale, di quanto ne abbia impiegato il Parlamento per approvarla. Ancora una volta l'irresponsabilità di parte della maggioranza aveva provato ad anteporre la cassaforte personale del Presidente del Consiglio alle tasche ormai vuote degli italiani, "salva-Fininvest" l'opposizione ha fatto, compatta, sbarramento, e devo dire anche qualche benpensante che pure continua ad esserci all'interno della maggioranza. Ma al senso dello Stato che l'Italia dei Valori ha mostrato venendo incontro alla preoccupazione degli italiani allarmati per il loro futuro, Libertà e la Lega hanno risposto con la consueta e per noi usuale arroganza, senza accogliere quasi nulla di quanto l'Italia dei Valori e le opposizioni hanno proposto. Ci sarebbe stato da mandare tutto all'aria, ma chi è pronto per la guida di questo Paese non ha inteso giocare al "tanto peggio, tanto meglio": agli interessi di parte ha voluto anteporre quello della nostra Italia. Dicevo che la manovra è pessima, senza equità, continua a privilegiare cassa e soliti furbi, per intenderci quelli che dopo l'*affaire* P4 si accingono a scaricare qualcuno per continuare a spartirsi la torta con la copertura di qualche altro. altro. Ministro Tremonti, il Governo di cui fa parte ha sempre negato con pervicace incoscienza l'esistenza della crisi manifestando un ottimismo di facciata. Più volte il Presidente del Consiglio, con esternazioni sempre più vuote (d'altra parte non ha avuto il coraggio di metterci la faccia neppure oggi) e per questo dannose, ha rivolto critiche alle opposizioni, le più variopinte: tristi, senza prospettive, cariche di odio. Ovviamente non era così, come purtroppo abbiamo sempre saputo, e penso se ne accorga anche egli stesso, se ogni tanto si guarda allo specchio. No, colleghi, nessuno dell'Italia dei Valori, con questo scenario, si è sentito di fare il bastian contrario; nessuno di noi voleva e vuole fare però la parte del fesso. In tre anni, tra manovre, manovrine, provvedimenti e leggine, ne avete approvate ben venti in materia finanziaria e di sviluppo, e di queste oltre la metà con il voto di fiducia. Le ultime settimane e questa manovra, signor Ministro, evidenziano il colossale fallimento della politica del Governo. La manovra è iniqua, non affronta nessun nodo strutturale, come pure l'Italia dei Valori ha richiesto da tempo e come da ultimo ha suggerito ancora ieri il Governatore della Banca d'Italia. Come al solito, la maggioranza è riuscita sempre meglio a centrare l'obiettivo che persegue dall'inizio della legislatura: togliere ai poveri e conservare privilegi e sprechi ai ricchi e ai potenti. Sui costi della politica non c'è nulla, e questa per l'Italia dei Valori è un'autentica vergogna. Nessun taglio delle indennità dei parlamentari e nessuna soppressione dei vitalizi; nessuna norma per l'accorpamento obbligatorio dei Comuni, per realizzare grossi risparmi; nessun taglio delle Province; nessuna cesoia sugli enti inutili, sugli stipendi supergonfiati dei *manager* pubblici; nessun aumento della tassazione delle rendite finanziarie; neppure le auto blu vengono toccate, e restano tutte le incompatibilità tra parlamentari e amministratori locali. Lei, a saldi invariati, ha cestinato ogni suggerimento che le abbiamo formulato, pur con le coperture necessarie. Questa manovra, Ministro, è un festival del non senso: altroché se mettete le mani nelle tasche degli italiani! I *ticket* sanitari partono immediatamente, senza distinzione di reddito: chi più ha chi più ha paga come chi nulla ha. Persiste, anche se impercettibilmente attenuato, l'odioso provvedimento contro le pensioni più basse, che vede permanere la tagliola delle rivalutazioni sulle pensioni. Ministro, dopo lo scudo fiscale che ha fatto lavare soldi oggetto di illeciti guadagni e di evasione fiscale con poco disturbo economico per i disonesti, oggi questa manovra schiaffeggia i contribuenti onesti: non quelli amici di Milanese, di Bisignani e della P4, ma quelli che hanno avuto il torto di pagare le imposte anche più del dovuto, e che non godranno né di rimborsi né di compensazioni. E che dire dei tagli lineari alle agevolazioni? Il Governo e la maggioranza colpiscono quelle sulla casa, quelle sulla famiglia, quelle su lavoro e pensioni, quelle per il terzo settore, quelle per le energie, rinnovabili le agevolazioni sanitarie, *handicap* compreso, le agevolazioni per le borse di studio: una platea di decine e decine di milioni di contribuenti. No, Ministro, così non va; se lei dichiara con una certa impudenza di stare bene al suo posto, gli italiani ben volentieri le restituirebbero il ruolo di cattedratico, lontano dal Ministero dell'economia e dalle tasche degli italiani. Liberalizzate senza liberalizzare, privatizzate senza regole certe, con il rischio che i gioielli dello Stato e società a capitale pubblico vadano sul mercato, facciano ricavare poco o niente (Alitalia *docet*) e arricchiscano speculatori o personaggi dall'incerto ed oscuro passato. Per questo, Ministro, noi speravamo speravamo che venissero introdotte norme serie per combattere l'evasione fiscale, ma ciò non è stato fatto. La Corte dei conti, ancora nei giorni scorsi, ha ribadito che questo grande salasso rappresenta un'ignominia per le casse pubbliche, come un'ignominia per le casse pubbliche è la corruzione pervasiva nella pubblica amministrazione. Noi francamente non abbiamo granché da sorridere, con questa manovra abbiamo dimostrato responsabilità di governo, mettendoci al servizio dei cittadini. Voi, che fino ad ora a nostro parere non lo avete fatto, a questo punto dovete rimettervi al giudizio dell'elettorato: abbiate questo coraggio, abbiate il coraggio di togliere le tende.

l'abbiamo ascoltata come sempre con grande attenzione e siamo lieti che lei abbia riconosciuto il ruolo delle opposizioni per tentare di mettere al riparo il Paese dagli attacchi speculativi sui mercati finanziari e, come lei ha ricordato nella sua relazione introduttiva, dalla sfiducia nei confronti dell'Europa, e purtroppo anche dell'Italia. Abbiamo chiesto noi di accelerare i tempi di esame e di approvazione della manovra, impegnandoci a non fare ostruzionismo, per consentire al Paese di dare in tempi rapidi una risposta istituzionale alla crisi di fiducia esplosa in queste settimane nei confronti dell'euro, in particolare con riferimento Tutto ciò l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente per il bene del Paese, grazie al Capo dello Stato. Con il dovuto rispetto, signor Ministro, non l'abbiamo fatto per lei, né per il suo Presidente del Consiglio, che da giorni si nasconde, non avendo il coraggio di spiegare al Parlamento e agli italiani perché ci troviamo in queste condizioni o di spiegare alla gente come si esce da questa situazione. Non l'abbiamo fatto per questa maggioranza irresponsabile, prigioniera di piccoli e grandi interessi corporativi che ingessano l'Italia impedendole di crescere. Non l'abbiamo fatto certamente in funzione di questa pessima manovra economica su cui chiedete la fiducia, una manovra iniqua e dannosa per le famiglie italiane e per i ceti più deboli, e che è la logica conseguenza, secondo noi, di tre anni di non governo che avete offerto al Paese: tre anni di *spot*, di promesse, di *slogan* populistici, di finte decisioni e di false riforme epocali, annunciate e mai realizzate. Oggi tutti i nodi vengono al pettine e siete costretti a fare una drastica manovra correttiva dei conti pubblici per riparare velocemente alle vostre manchevolezze e alla vostra strutturale incapacità politica di governare il Paese. Nel luglio 2009, signor Ministro, illustrando la finanziaria qui in Senato, lei ebbe modo di affermare che in caso di maggiori entrate vi sarebbero stati possibili interventi per le priorità più urgenti e che ci saremmo dovuti aspettare un rimbalzo positivo entro il 2010. Quel rimbalzo lo stiamo ancora aspettando. A settembre dello stesso anno, il suo Presidente del Consiglio accusò le opposizioni di essere anti italiane,

L'uscita dalla crisi la stiamo ancora aspettando, e oggi, in un momento particolarmente difficile per l'Italia, se non ci fosse stato il Presidente della Repubblica e queste opposizioni responsabili, sareste a «Chi l'ha visto?» in cerca del Presidente del Consiglio che, come sempre, ha paura di assumersi le sue responsabilità. Ancora l'11 marzo del 2010, il suo Primo Ministro annunciava che grazie a Tremonti i conti pubblici sono sotto controllo, che «la crisi è alle spalle, è iniziata la risalita, ma è lenta». Quanta acqua è passata sotto i ponti, signor Ministro, anche nei suoi rapporti con l'onorevole Berlusconi, a quanto - ahinoi! - leggiamo sui giornali? Per carità di Patria mi fermo e non proseguo nelle citazioni che riguardano lei e il presidente Berlusconi, e i tanti, troppi Ministri del suo Governo, improvvisati «Harry Potter» della politica, pronti a dichiarare che l'Italia è grosso modo il Paese del Bengodi. Certo non sarà sfuggita neanche a lei una delle ultime dichiarazioni del presidente Berlusconi, che mi pare risalga al 23 dicembre scorso: una manovra correttiva perché non c'è né la previsione né la necessità». E invece oggi siamo qui, di fronte alla responsabilità di azzerare il *deficit* entro il 2014, e di dover trovare per quella data oltre 40 miliardi di euro, se vogliamo stare in Europa, che rischiano comunque di non bastare, come appena ieri ci ricordava il Governatore della Banca d'Italia. In un Paese come il nostro, che non cresce perché non avete voluto fare, e non farete mai, le liberalizzazioni e le privatizzazioni, oltre alle cosiddette riforme strutturali nel settore della pubblica amministrazione, dello Stato sociale e del fisco, in preda a una in preda a una profonda e permanente crisi politica e di credibilità interna ed internazionale del Governo e della maggioranza, vi presentate in Parlamento con una manovra - non me ne voglia, signor Ministro - degna dei tanti Ministri e dei tanti Governi della Prima Repubblica, che non taglia efficacemente la spesa e che aumenta le tasse. Sì, signor Ministro, continuate a far mettere le tasse alle Regioni e agli enti locali, a cui tagliate ancora una volta i trasferimenti. Ed ora avete cominciato a metterle direttamente voi, le mani nelle tasche degli italiani, con il *ticket* sulle prestazioni sanitarie, che avete pure inasprito in queste ore, senza alcuna considerazione per le famiglie più disagiate. Incidete profondamente su pensioni e risparmi, dopo aver detto per anni che non c'era la necessità di riformare le pensioni e che mai avreste introdotto una patrimoniale. Avete fatto l'una e l'altra cosa e, se non fosse stato per noi, per gli emendamenti, che insieme ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori abbiamo presentato, lo avreste fatto in maniera ancora più selvaggia, in danno delle famiglie italiane e dei piccoli risparmiatori. Siccome tutto ciò non basta, siete costretti a fare una riforma fiscale che prevede da 15 a 20 miliardi di maggiori entrate. Questa manovra è la prova evidente del fallimento del Governo e della politica del centrodestra. Mette fine alle vostre parole d'ordine: federalismo (perché resta in vita solo quello delle tasse); taglio delle tasse (ne prevedete circa 30 miliardi in più); libertà economiche (grazie al partito degli avvocati e dei monopolisti pubblici e privati che vi comandano, lei, signor Ministro, si è rimangiato in tempo reale la norma che ci mette in linea con l'Europa). Questa manovra non ci piace perché non aiuta la crescita e lo sviluppo, perché non dà una voce di speranza al Sud e, anzi, persevera nell'accanimento leghista contro le aree più deboli del Paese. Senza crescita e senza sviluppo non si tengono i conti in ordine. Potete continuare a tagliare e a tassare il Paese, ma la situazione non cambia. Un Paese che spende più di quanto guadagna ha bisogno di far crescere la ricchezza e di ridurre il debito pubblico: voi non fate né l'una né l'altra cosa. Siamo certamente d'accordo con la sua proposta relativa al pareggio di bilancio, ma, come lei sa, essendo una modifica costituzionale, ha bisogno di almeno due anni. Dal 2001 ad oggi, anche a causa del finto federalismo, la spesa pubblica è passata dal 48 per cento del prodotto interno lordo al 51 per cento. Il nostro debito è pari al 120 per cento del PIL, esattamente il doppio degli americani. La pressione fiscale è aumentata, e la crescita economica non si vede. Non è con risposte pavide dal punto di vista politico che si governa il Paese, signor Ministro - e non faccio un torto a lei, ma a ciò che rappresenta la sua maggioranza magari di scaricare sui vostri successori l'onere della impopolarità, impegnando così pesantemente per il risanamento dei conti i primi due anni della prossima legislatura. Tra l'altro, lo fate anche in malafede, tanto da introdurre in questa manovra la cosiddetta clausola di salvaguardia, che prevede un taglio lineare del 15 per cento di tutte le agevolazioni fiscali per coprire un eventuale e prematuro buco di bilancio. Sì, risposte pavide, come quelle sui costi della politica, il cui contenimento volete per gli altri e non per noi, come per le Province, rispetto a cui non avete voluto accogliere neanche un nostro emendamento di buon senso e mediazione che prevedeva l'accorpamento di quelle con meno di 500.000 abitanti, o per i piccoli Comuni, per i quali abbiamo proposto l'accorpamento, almeno per quelli fino a mille abitanti, nella convinzione che solo così possono essere mantenuti in vita e li si può promuovere, altrimenti moriranno per consunzione, non avendo né ricchezza propria né trasferimenti erariali. anche per le incompatibilità tra l'incarico di sindaco e di parlamentare, di consigliere regionale e di consigliere provinciale, di doppi e tripli incarichi. Di tutto questo però a voi non interessa nulla. Vi lavate la coscienza con interventi modesti sui voli di Stato e le auto blu - per i quali, comunque, viste le ristrettezze economiche, non potremo più pagare neanche la benzina e la manutenzione senza intervenire sui veri costi della politica, quelli che paga veramente il Paese, che sono gli sperperi delle tante zone grigie del Paese e la corruzione. Potete continuare a dire che è colpa degli altri, a partire dall'euro e dagli speculatori, ma non è così, o meglio, non è solo o meglio, non è solo così. Non potete però continuare a nascondere che una parte importante del problema siete voi: è questo Governo, è questa maggioranza debole, confusa e litigiosa che mostra in pubblico la mancanza di fiducia del Presidente del Consiglio nei confronti del più importante dei suoi Ministri, quello dell'economia. *(Applausi del senatore Peterlini).* unita all'assenza di una visione strategica del futuro dell'Italia, vi impongono un gesto di responsabilità, pari se non superiore al nostro: passare la mano, per adottare insieme gli interventi importanti che servono al Paese. Quegli interventi che voi da soli non sapete, non volete e non potete fare. Per queste ragioni, vi diciamo ancora una volta: no! Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, abbiamo vissuto una settimana particolarmente intensa, a tanti di noi sono venuti un bel po' di capelli bianchi in più. Tuttavia, la reazione del Governo, del Parlamento, delle istituzioni è stata molto forte, straordinaria, o meglio straordinaria e normale al tempo stesso. Straordinaria, perché si giunge ad approvare una manovra che ci fa raggiungere per davvero il pareggio di bilancio nel 2014, operazione che è riuscita a questo Paese una volta sola due secoli fa, in soli tre giorni, quando di solito per approvare una manovra impieghiamo tre o quattro settimane. Straordinaria, anche perché la manovra è stata potenziata e irrobustita molto dal punto di vista dei saldi e notevolmente migliorata nei punti critici, condivisi anche dall'opposizione e con l'opposizione: le pensioni, la tassa sui depositi, il patto di stabilità, gli investimenti in infrastrutture.

sui pochi emendamenti da presentare (la Lega Nord ne ha presentati solo cinque, sui cinque temi che andavano messi a posto). Questo è un patrimonio importante; però, non possiamo illuderci che i problemi siano già tutti risolti. In particolare, resta il problema dell'euro e dell'Europa. È chiaro il rischio che il nostro Paese corre in caso di attacchi sul fronte del debito, attacchi che si estendono anche ai nostri principali istituti bancari.

anche se dall'opposizione viene una critica, in particolare, su quei 20 miliardi, soldi veri, derivanti dalla delega sul riordino delle agevolazioni fiscali. Al riguardo, vi riporto una citazione testuale: «Giusto è invece il progetto di diradare la foresta delle detrazioni. Molte di queste sono del tutto ingiustificate e non servono in alcun modo alla crescita dell'economia.

questo passaggio perché quando si affrontano i temi nel concreto, le soluzioni poi non hanno colore politico. Infine, ricordo i contributi della Lega Nord alla manovra. Sulle pensioni: nessun blocco alle più basse, recuperando soldi dal taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Sull'imposta sul deposito titoli si tutelano i piccoli risparmiatori.

In ultimo, il patto di stabilità. Da un lato - e questo è molto importante - si rende operativo da subito l'obbligo di accorpare le funzioni dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che sono la stragrande maggioranza. Da questo obbligo è evidente a tutti che si ricaveranno ingenti e importanti risparmi. Dall'altro, si fissa il principio per cui i tagli non saranno più uguali per tutti:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questa manovra non è la nostra. Ne contestiamo l'impostazione ed i contenuti e non la voteremo. È, credo, il dodicesimo provvedimento economico di questo Governo in tre anni, l'ennesimo negli ultimi 10 anni in cui, quasi ininterrottamente salvo i 20 mesi del secondo Governo Prodi, avete governato questo Paese. Tralascio la *querelle* tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia che ha accompagnato la genesi di questa manovra finanziaria. Ricordo, però, che sin dall'inizio vi dicemmo che mancavano 15 miliardi. Avevamo ragione noi. E se oggi ci avviciniamo a quell'obiettivo di rafforzamento della ci raccomanda, e ci avviciniamo accorciando un po' le distanze all'obiettivo del pareggio di bilancio, è perché quella obiezione è stata fatta e con tanta determinazione sostenuta. Vi abbiamo chiesto più equità, più regole e più crescita. Avete dato troppo poco. Avete accentuato l'iniquità di questa manovra con i tagli del 20 per cento ai presidi essenziali del *welfare.* Vede, senatore Garavaglia, certo che ci sono - come dice il ministro Tremonti - 480 meccanismi di detrazione fiscale.

E se si anticipa l'entrata in vigore del *ticket* sulla diagnostica ambulatoriale il risultato è che non si agevola il pubblico ma il privato, e questo ovviamente speculando sul diritto alla salute. Vi abbiamo proposto norme che mettessero ordine nel bilancio. E avete detto no. Vi abbiamo chiesto delle liberalizzazioni che potevano farsi subito. E ci avete detto no seppure questo delle liberalizzazioni sia uno dei capitoli sui quali l'Europa ha attirato l'attenzione ha sottolineato l'importanza, anche negli ultimi recenti colloqui che lei ha avuto in quella sede. Chiedete sacrifici agli italiani e non siete stati capaci di fare quattro cose che vi avevamo chiesto: chiesto: allineare le retribuzioni dei parlamentari al parametro europeo, ancorare i vitalizi parlamentari al criterio contributivo, tassare le pensioni dei parlamentari allo stesso modo con cui vengono tassate le altre pensioni d'oro, e riordinare il sistema delle Province. Erano quattro cose che sono state oggetto dei nostri emendamenti e di cui non c'è traccia Vi avevamo proposto un piano industriale della pubblica amministrazione che riorganizzasse gli uffici periferici, recuperando risorse ed efficienza. E ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto più regole e ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto alcune misure per la crescita. Ovviamente avete detto no. Vi avevamo proposto anche una soluzione moderna per la internazionalizzazione delle imprese. Avete risposto con una burocratizzazione

però, impedirla, e tutte le volte in cui in questi tre anni vi siete rifiutati di rimuovere con legge gli ostacoli strutturali alla crescita, voi avete mancato l'obiettivo. Mentre in qualunque Paese, in queste circostanze, il Capo del Governo sarebbe stato in contatto diretto e continuo con il Parlamento, con i suoi Ministri, con la Banca d'Italia, con l'Europa e con i circoli finanziari, il vostro Presidente del Consiglio è rimasto chiuso nella sua cassaforte, come Paperon de' Paperoni, abbracciato al sacco dei dobloni piangendo perché glieli stavano portando via. Fuori infuriava la tempesta e voi eravate, ovviamente, paralizzati dalla paura e stavate paralizzando il Paese, preoccupati assai - e mi pare con ragione

Non siete stati all'altezza e non avete avuto il coraggio. Mentre questo accadeva e sull'Italia si scatenava non solo il rischio, ma la realtà di una furiosa manovra speculativa - lasciatemelo dire, colleghi della maggioranza - voi annaspavate. Lì abbiamo capito che c'era una sola cosa da fare: opporre ai nemici dell'Italia semplicemente l'Italia, non un Governo in difficoltà, non una maggioranza divisa e frastornata (ragioni prime della debolezza dell'Italia sui mercati finanziari), non un'opposizione sociale oltre che politica, santamente inferocita, ma l'Italia intera e unita: l'Italia di Giorgio Napolitano. Abbiamo avuto il privilegio di poterlo fare perché apparteniamo all'Italia essendo, oggi, il più grande Partito italiano l'onore e la responsabilità di rappresentarlo. È un Partito che è il caleidoscopio di tutto il Paese da ogni punto di vista (sociale, demografico, territoriale, economico e generazionale). Lo abbiamo potuto fare perché qui al Senato - lo dico perché sono il Presidente del Gruppo del Senato - abbiamo un Gruppo parlamentare di prim'ordine. *(Commenti Lo dico perché mentre voi litigavate fra di voi, questo Gruppo parlamentare, conoscendo il costo politico di rinunciare a emendamenti e pretese, ha dato una prova di responsabilità che non siete capaci di sognarvi. Ma non siamo stati soli. Questo è un fatto politico di primo rilievo:

La nostra scelta è stata autonoma, perché non ce l'avete chiesto. Casomai, devo ringraziare il presidente Schifani di aver accolto con tempestività la nostra tempestiva scelta coraggiosa, anche rispetto ai nostri elettori, e responsabile. Lo abbiamo fatto per l'Italia e non per voi. Abbiamo dato un contributo un contributo serio a spegnere l'aggressione speculativa nei confronti del Paese. Non è un merito che ci attribuiamo da soli, ma che ci riconoscono commentatori italiani ed europei. L'unico che non lo dice è il presidente Berlusconi, ma francamente ce ne infischiamo. Non a questo Governo dobbiamo rendere conto. Mentre le opposizioni presentavano solo 25 emendamenti, voi presentavate un maxiemendamento solo

notizia. Se l'Italia avrà entro la settimana la manovra approvata, sia pure con tutti i limiti e i difetti che vediamo e denunciamo, se l'Italia sarà più forte, io qui ne rivendico il merito all'opposizione. Non siete stati di capace di cogliere l'occasione. Ancora una volta vi sono mancati il cuore e la generosità, che, secondo me che sono dirigente politica donna, sono categorie della politica.

di fronte all'Italia di dimettervi. Il vostro Governo è un danno per l'Italia. Un grande Paese che può farcela assai meglio senza di voi.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori,

Quindi, è difficile subire lezioni. Ma non voglio alimentare eccessive polemiche, anche se qualcosa dovrò dire perché rivendico al nostro Gruppo (131 senatori) e alla maggioranza di aver concentrato in cinque proposte emendative la nostra azione e di avere per primi chiesto l'accelerazione dei tempi parlamentari. Una settimana fa, il 6 luglio, il segretario del Partito Democratico diceva di cambiare il decreto che stiamo discutendo in un disegno di legge, garantendone l'approvazione entro il 30 settembre. Apprezziamo che ci sia stato un mutamento di idee, consapevoli dei problemi che l'economia internazionale sta vivendo, e ve ne diamo atto volentieri. È una crisi dell'euro, una crisi dell'Europa. Ha detto nei giorni scorsi Jean-Paul Fitoussi: «Gli aiuti alla Grecia sono arrivati tardi e intanto la speculazione ha continuato ad operare, anzi si è convinta che poteva attaccare più in alto della Grecia: Portogallo, Spagna, Italia e forse Francia o Germania. Il fatto che una vicenda piccola della Grecia abbia causato questa crisi spaventosa dimostra la debolezza politica dell'Europa ed è un peccato imperdonabile, vista la ricchezza potenziale del continente. I mercati» - dice Fitoussi - «hanno messo l'Europa sotto tutela perché la politica europea lo ha consentito. La colpa è dell'Europa che si sta dimostrando solo un'espressione geografica. Bisogna rilanciare il disegno europeo». Nei giorni scorsi, Romano Prodi, che ha guidato l'Europa per alcuni anni ed al quale non vogliamo attribuire colpe esclusive, ha detto che l'Europa ha pesantemente fallito. Beh, faccia anche lui qualche riflessione autocritica

Nel Congresso americano si sta discutendo della possibilità che ci sia un *default*, che in italiano vuol dire fallimento, dell'economia americana; e poiché Obama, che noi rispettiamo e voi osannate, non ha più la maggioranza in uno dei due rami del Parlamento, deve negoziare con i repubblicani se aumentare le tasse o tagliare le spese, per un piano di 4.000 miliardi di dollari in 10 anni. Negli Stati Uniti d'America ildeficit ha infatti raggiunto il valore del PIL e se non ci sarà un accordo entro il 2 agosto - e non ce lo auguriamo, perché siamo tutti collegati, non solo nell'euro, siamo tutti in una comunità internazionale - il fallimento si verificherà. Questo è il mondo in cui oggi stiamo governando: governiamo al tempo della crisi con proposte all'altezza dell'interesse del nostro Paese. Questo è il nostro impegno. Vogliamo parlare delle speculazioni sui mercati internazionali e della concorrenza sleale che alcune parti del pianeta fanno all'Italia e all'Europa? C'è uno scontro tra piattaforme continentali. Lo sapete che le riserve valutarie della Cina sono aumentate del 30 per cento rispetto allo scorso anno e che la Cina ha un tesoro di 3.200 miliardi di dollari; si tratta di una cifra astronomica, mai raggiunta prima nella storia dell'economia mondiale. Ma ciò che fa ancora più impressione è che continua a crescere e che in dieci anni le riserve della superpotenza asiatica si sono moltiplicate per 18 volte. A tutto questo opponiamo un sistema che ha la sua solidità: Il tanto citato governatore della Banca d'Italia, Draghi, ieri, all'assemblea dell'ABI, ha detto che dopo sei mesi di variazioni appena positive, nel secondo trimestre il prodotto interno dell'Italia è cresciuto ad un tasso in linea con quello medio dell'area dell'euro, che la manovra del Governo rappresenta un passo importante per il risanamento dei conti pubblici, che quest'anno ci sarà un surplus primario significativo e che l'anno prossimo crescerà ancora. Parla Draghi e i riconoscimenti sono alla politica di questo Governo e alla politica che in queste ore stiamo discutendo. Questa manovra razionalizza la spesa delle amministrazioni pubbliche, interviene in maniera cauta, senza alcuna macelleria sociale, sui temi della previdenza dal Gruppo PD)* con interventi graduali che servono a garantire il futuro delle pensioni dei nostri figli, perché senza interventi distruggeremmo il sistema previdenziale e compiremmo un attentato verso le nuove generazioni! Si introduce una fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, si prevede la soppressione e il riordino di molti enti e organismi pubblici, si interviene sulla banda larga, sul rifinanziamento del fondo infrastrutture. Il nostro Gruppo è intervenuto con pochi emendamenti per rendere più equa l'azione sulle pensioni, per tutelare le fasce più basse, basse, per rendere più equo l'intervento sul risparmio e per tutelare il piccolo risparmio e per garantire gli investimenti nelle opere pubbliche, correggendo la norma sugli ammortamenti. Siamo intervenuti anche affinché si modificasse il Patto di stabilità. Stiamo attenti a tutte le aree del Paese, ma non dimentichiamo che

abbiamo ritenuto di sostenere - e lo affermiamo anche in Parlamento - che i processi di liberalizzazione vanno portati avanti, senza però mettere a repentaglio una ricchezza di competenze e professionalità tutelata dall'articolo 33 della Costituzione! Difenderemo sempre competenze e professionalità accanto ai processi di liberalizzazione nel nostro Paese. Abbiamo affrontato con immediatezza la situazione, chiedendo tempi rapidi e diamo atto a tutti di avere condiviso queste procedure. Desideriamo ringraziare in maniera non formale il Presidente del Senato per l'equilibrio, la saggezza con cui ha seguito

degli obiettivi indicati. Voglio ancora ringraziare il presidente Azzollini, il relatore Pichetto Fratin, i sottosegretari Giorgetti e Gentile, il ministro Tremonti e tutto il nostro Gruppo, che come qualità, competenze e serietà ha dimostrato ancora una volta di essere il primo Gruppo del Parlamento

italiana. Volete governare in futuro? Vi attenderemo alla prova (non credo che accadrà), per sapere cosa farete sui trasporti, sulla TAV, sull'energia, sulle municipalizzate. A proposito di costi della politica, in questi anni di Governo del centrodestra abbiamo ridotto del 30

Avevamo approvato anche una legge sui servizi pubblici locali che tagliava le mani ai partiti sul territorio; oggi tutti parlano di privatizzare, di aprire al mercato queste realtà. Noi lo avevamo fatto e voi avete sostenuto un *referendum* che ha ridato il potere alla partitocrazia sui territori! Questa è la verità! Nel 2006, con un altro *referendum,* avete impedito alla nostra proposta, che non fu confermata a livello popolare, di ridurre il numero dei parlamentari. Gli effetti dal Gruppo PdL).* Meno *referendum* a favore dei partiti e delle poltrone, più leggi per ridurre davvero i costi della politica e dei tanti apparati pubblici finanziati con soldi pubblici. Anche su questo terreno non temiamo la sfida, ma la raccogliamo: abbiamo realizzato fatti ed in questa

e ci auguriamo di poter credere, signor Ministro, anche nell'Europa di cui lei ha parlato con realismo. Non siamo euroscettici e faremo la nostra parte per non diventare eurodelusi. Difendere i conti pubblici vuol dire difendere le fasce più deboli della popolazione, difendere gli anziani e i nostri figli, difendere le pensioni e gli ammortizzatori sociali. Dobbiamo quindi assumerci la responsabilità di questa manovra; lo facciamo di fronte al Paese prendendo atto delle collaborazioni e respingendo le critiche. Oggi, con questo voto di fiducia, si confermerà la saldezza di questo Governo che continuerà ad andare avanti perché l'Italia cresca, perché l'Italia viva.

nell'esprimere soddisfazione e condivisione per la funzione di guida svolta dal Presidente della Repubblica a fronte delle drammatiche condizioni finanziarie in cui versa il Paese, nel condividere altresì l'appello alto rivolto dal presidente Romano Prodi dalle colonne de «Il Sole 24 Ore», a nome del Partito repubblicano italiano esprimo apprezzamento per i provvedimenti di taglio di spesa contenuti nella manovra, che consideriamo inevitabili per l'aggiustamento dei conti, sebbene ancora scarsamente finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico, ma indispensabili comunque per bloccare la speculazione finanziaria internazionale. Il rigore di oggi, ministro Tremonti, assicura il domani per i nostri figli. Confidiamo pertanto nella sua seria volontà di proseguire nell'opera di risanamento dei conti pubblici e di pareggio di bilancio e la incoraggiamo a continuare nel suo difficile lavoro per il bene del Paese. Come repubblicana, comunque, con il senso di responsabilità che mi impone, oltre che la mia storia, la gravità della situazione del Paese, nel dare l'assenso alla manovra e nell'assicurare che i repubblicani manterranno una vigile attenzione rispetto all'attuazione dei provvedimenti in essa contenuti, per una mia personale coerenza rispetto alla fiducia richiesta, dichiaro di non partecipare al voto.

la Presidenza non poteva che prendere atto delle osservazioni svolte dal Presidente della 5a Commissione a conclusione della riunione. Il presidente Azzollini ha ricordato infatti come, nonostante le criticità di natura finanziaria indicate dall'opposizione, il Governo abbia invece affermato che la norma è provvista di copertura con le argomentazioni poc'anzi illustrate. I precedenti della XIV e della XV legislatura a cui il senatore Morando ha fatto riferimento vanno ricondotti a casi in cui la Commissione bilancio aveva riscontrato problemi di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla questione però - e ciò naturalmente non può che farmi piacere - ha chiesto di intervenire il ministro Tremonti. Onorevoli

Signor Presidente, onorevoli senatori, senatore Morando, lei ha rappresentato un caso che ha certamente una consistenza, ma - se mi permette il rilievo - non ha la consistenza materiale che lei ha rappresentato. Io credo che, comparando quanto vi sarebbe di ingiusto eliminando quella norma e quanto comunque di positivo per l'economia e, di riflesso, anche per il bilancio pubblico,

presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.